del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*** gli articoli 5 e 6 ha avuto inizio l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 e dei subemendamenti all'emendamento 7.900 del Governo. Il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario su tutti gli emendamenti e i subemendamenti, ad eccezione dell'emendamento 7.900.

Su richiesta di un Gruppo parlamentare, la Presidenza ha accordato una sospensione dei lavori fino alle ore 10,30. Sospendo pertanto

Il Senato è in numero legale.

però quanti emendamenti vengono accorpati. Almeno questa prassi mi sembrava che si fosse instaurata. Se si decide di applicare il canguro, almeno si mettano i senatori nella condizione di sapere, prima del voto che poi preclude tutti gli altri emendamenti, quanti altri emendamenti vengono preclusi. Avete contingentato i tempi, avete mortificato il confronto, siete rimasti in silenzio per tutto il tempo, almeno spiegateci com'è che volete applicare questo canguro. È una vergogna!

Presidente, devo dire che, dopo la giornata di ieri, soprattutto per quello che è successo alla Camera dei deputati, mi sarei aspettata un atteggiamento diverso per questa ultima parte del nostro dibattito, quantomeno che si potesse articolare meglio e lasciare alle opposizioni lo spazio

prosieguo di dibattito speriamo di poterlo fare in modo puntuale e in modo tale che non sia semplicemente un lavoro di ostruzionismo, che pure è legittimo, in quanto noi vogliamo poter articolare in modo puntuale le nostre posizioni.

Noi sappiamo come sia difficile lavorare quando il clima non è positivo; come sia difficile lavorare e provare a dibattere quando sappiamo esattamente che non c'è interesse da parte degli altri. Quelli che stiamo provando a fare sono interventi nel merito e cercano di ristabilire un po' di armonia,

ha provato anche ieri a sollecitare il dibattito in un clima non positivo e non di ascolto. Noi continuiamo a ribadire la necessità che quei tempi che ci sono stati tagliati, dopo che

facendo è un lavoro che la maggioranza ci dice che vuole svilire; non posso credere che i colleghi vogliano svilire il lavoro dell'opposizione. Al netto di quelli che possono essere le diatribe e i dibattiti, voglio riconoscere alla maggioranza la capacità di cogliere la necessità che l'opposizione abbia voce; sono convinta che la maggioranza e la Presidenza condividano questa necessità. Rivedete quindi le posizioni.

Signor Presidente, noi non smetteremo di illustrare le ragioni della nostra forte contrarietà a questa riforma anche in pochi secondi, anche in un minuto, perché abbiamo rispetto delle istituzioni e lo facciamo di fronte ad una maggioranza silente e che fa fatica a mantenere il numero legale. *(Applausi)*. Per noi il Parlamento è l'espressione più alta della democrazia rappresentativa; è il luogo dove si prendono le decisioni a favore dei cittadini e del Paese. Non possiamo accettare che nel silenzio e nella mancanza di argomenti, con un atteggiamento assolutamente di sudditanza nei confronti del Presidente del Consiglio, il Parlamento venga svilito. Continueremo a dirvelo oggi e nei prossimi giorni, perché questa è una battaglia a favore della nostra Costituzione.

Signor Presidente, ieri abbiamo posto una domanda di merito seria. Vorremmo che la maggioranza prendesse la parola e ci dicesse per quale ragione bisogna differenziare la disciplina degli effetti della interruzione del rapporto di fiducia, a seconda che tale interruzione avvenga a seguito di una mozione di sfiducia, oppure a seguito di un voto contrario delle Camere su una questione di fiducia posta dal Governo. È una questione seria, non non un intervento capzioso. Qualcuno della maggioranza prenda sul serio questa nostra considerazione e risponda nel merito. Questa distinzione che oggi il testo prevede a noi risulta del tutto incomprensibile.

Signor Presidente, per il suo tramite mi rivolgo ai colleghi della maggioranza e anche alla Ministra, che ha avuto

Non è così che si fanno le riforme che servono a un Paese. Non è così che si tutela la governabilità e quello che fate oggi potrebbe domani risultare enormemente dannoso, anche quando voi sarete all'opposizione. Non si fanno mai le riforme pensando solo al proprio interesse. Dentro a questa riforma esce fuori soltanto questo: voi pensate di rimanere al Governo per sempre. Non sarà così, perché la democrazia, per fortuna... Signor Presidente, devo dire che un po' mi sconcerta l'atteggiamento remissivo e quieto di quest'Assemblea, dopo quanto è accaduto ieri. Stiamo facendo le prove per il bavaglio ai parlamentari, per la remissività e l'essere chini al potente di turno in un clima da atteggiamento davvero di silenzio e remissione. Vorrei usare dei termini che verrebbero sicuramente censurati dal Presidente, ma devo dire che gli attacchi squadristi e fascisti visti ieri alla Camera dei deputati *(Applausi)* nei confronti del nostro collega Donno

parlamentari completamente silenti, abbiamo una schiera di "signorsì signore", che non pensano con la propria testa e che semplicemente votano a comando.

la trattazione di questo provvedimento è fatta in modo delegato e autoritario. Il Governo ha detto "fate così" e la schiera dei parlamentari della destra al Governo è una schiera di "signorsì signore" ed è una questione indecente. Il contenuto di questa riforma è pericolosissimo, è drammaticamente pericoloso per la democrazia italiana. È un provvedimento che, sia nel merito sia nelle forme, sta per essere licenziato in modo autoritario, senza cervello, senza la testa dei parlamentari che lo stanno approvando. Questa deriva autoritaria non sta solo negli atti, ma sta pure nei fatti, perché quello che è accaduto ieri è un fatto di gravissima violenza fisica che rappresenta che cosa stia nella testa dei parlamentari di maggioranza. Siamo in Italia, siamo nel 2024,

Mi faccia dire che il modo in cui stiamo discutendo queste riforme da questo lato del Parlamento, ma anche dall'altro della Camera, è davvero deprimente rispetto alla forza, invece, che un dibattito parlamentare di riforme di tale portata dovrebbe avere. Si è parlato di rissa, ma quello che è successo ieri è stata un'aggressione alla Camera dei deputati. C'è un clima di non ascolto, c'è un clima pessimo rispetto a quello che è davvero in discussione. che noi siamo per rimettere al centro il Parlamento, i suoi poteri e la possibilità che in Parlamento si risolvano le crisi e quindi si dia mandato a un'altra persona - come dice questo emendamento

nel dichiarare il voto contrario su questo emendamento, vorrei intervenire a difesa della dignità dei parlamentari. La dignità del dibattito consiste anche nel non dire menzogne, non continuare a dire che la maggioranza non è mai intervenuta, perché è intervenuta, sia pure quasi sempre (se non sempre) tra gesti,

In secondo luogo, luogo, auspicherei - e mi appello, per suo tramite, al Presidente - che si smettesse di accusare gli altri di essere senza testa, burattini,

Viene continuamente detto dall'opposizione che, siccome una sfiducia nei confronti del Governo può portare a dimissioni del Governo e dunque ad elezioni anticipate, i parlamentari sono legati, sono al guinzaglio, sono burattini e via dicendo. che non è così; almeno, se qualcuno ragiona in questo modo, ossia se pur di stare qui continua a votare per il Governo, anche se in quel Governo non ha più fiducia, allora è vero. Ma se chi pensa che il Governo debba andare a casa per il bene della Nazione e vota contro il Governo o non vota la fiducia, allora non è più così.

sarebbe stato sufficiente che i deputati e i senatori continuassero a votare la fiducia al Governo per non andare a elezioni anticipate; invece i deputati e i senatori dell'epoca - forse hanno fatto bene, forse hanno fatto male - scelsero liberamente di non dare la fiducia a quel Governo e si andò a elezioni anticipate, cosa che accadde ancora nel 1983,

Nella scorsa legislatura, ad agosto 2019, il primo Governo presieduto da Giuseppe Conte non ha più avuto la fiducia; sarebbe bastato continuare a dargli la fiducia e si sarebbe andati tranquillamente fino a fine legislatura, cosa che poi è avvenuta ma in modo del tutto imprevedibile,

perché due dei Gruppi che lo sostenevano non lo sostenevano più, sapendo bene che si sarebbe andati ad elezioni anticipate. Dunque non gettate fango sulla dignità dei parlamentari perché i parlamentari sono capaci di affrontare le elezioni. *(Applausi)*. Perché in democrazia le elezioni non sono una disgrazia. Bisognerebbe poi rispettare il mandato degli elettori, che è ciò a cui questa riforma mira.

È pacifico che una maggioranza parlamentare possa, in qualunque momento, decidere il proprio scioglimento. Il punto è se possa anche decidere soltanto di dimissionare il Governo, senza per forza essere...

Credo che lei lo sappia bene. Pertanto, a proposito di dignità dell'argomento che viene usato, lei fa torto all'intelligenza dei nostri colleghi se pensa che non sappiano la differenza tra l'autoscioglimento, quando la maggioranza ritiene che non ci siano più le condizioni politiche per dare vita a un Governo, e quando...

consentire al *Premier* eletto, anche qualora non raggiunga la fiducia, laddove la pone, di continuare ad andare avanti. Quindi i parlamentari non hanno alcuna arma per dire al Governo che non ha più la loro fiducia. Il *Premier* eletto può andare avanti comunque, in ogni circostanza, eccetto quando decide di dimettersi, e in quel caso muore anche il Parlamento. Quindi, quello che lei afferma è falso, altrimenti avreste approvato il cosiddetto emendamento Pera. Inoltre, la vostra difesa del Parlamento e della democrazia perde di ogni credibilità nel momento in cui in quest'Aula non ho ancora sentito una voce di condanna da parte della maggioranza per l'aggressione fascista avvenuta ieri alla Camera dei deputati. *(Applausi)*. Non siete credibili. Credere, obbedire, combattere: questo è il vostro motto.

il presidente Malan ha delle ricostruzioni abbastanza fantasiose. Rivolta sempre il calzino, a seconda di come conviene. È normale, in quanto è il ruolo che gli compete in maggioranza.

cosa significa che non si toccano i poteri del Presidente della Repubblica se adesso può decidere di affidare l'incarico di formare un nuovo Governo a chi è in grado di formare una nuova maggioranza e, invece, con il vostro disegno,

volevo, per suo tramite, fare una chiosa sulle parole del senatore Malan, al quale volevo ricordare che si getta fango sul Parlamento anche con gesti e affermazioni che lo disonorano. E sarebbe bene che anche da quest'Aula venisse una condanna forte dei gesti e delle affermazioni che disonorano il Parlamento.

Il 13 giugno 1944, esattamente ottanta anni fa, più o meno in queste ore, a Forno, un borgo apuano del comune di Massa

Nel momento in cui viene applicato il Regolamento e viene concesso un minuto in più, le urla in questo modo io non le accetto. Lo dico a lei, perché è quello che ha urlato di più, ma lo ricordo a tutti. *(Applausi)*. Non mi interessa essere applaudito. Sto concedendo un minuto in più, Sto concedendo un minuto in più, ma, nel momento in cui il minuto è terminato, si passa alla votazione.

martedì alle 15,30 avranno inizio le dichiarazioni di voto, anche se poi non è stata votata la vostra richiesta di modifica del calendario, in realtà, rispetto al tempo che era stato concesso rappresenta di fatto un favore che viene fatto all'opposizione. Questo perché, ore i tempi che rimanevano, fondamentalmente avremmo chiuso il provvedimento e saremmo arrivati alla fine dell'esame degli emendamenti: perché questo era previsto ed era stabilito con il tempo a vostra disposizione. Il fatto di fissare a martedì prossimo alle 15,30 l'inizio delle dichiarazioni di voto ha, nel concreto, dato la possibilità alla minoranza di usufruire delle ore della giornata di oggi e anche delle eventuali ore stabilite nella giornata di martedì, che

stabilendo che martedì alle 15,30 inizieranno le dichiarazioni di voto, è evidente che, in base alla programmazione dei lavori, noi dobbiamo finire di votare gli emendamenti. Se ogni Gruppo continua, ad ogni emendamento, a fare una dichiarazione di voto di un minuto, perché questo è previsto dal Regolamento, noi andremo avanti una settimana.

e quindi andiamo avanti tre settimane che stiamo discutendo in Aula di questo provvedimento, quindi non è che non stiamo discutendo. Si può essere favorevoli o contrari, ma veniamo incontro a quello che è un *gentleman agreement* che è già stato stabilito e che ci ha visti protagonisti, al di là delle singole posizioni, nella Conferenza dei Capigruppo.

la nostra disponibilità c'è stata, se poi dall'altra parte c'è il muro contro muro, vorrà dire giustamente che si agisce secondo il Regolamento. Presidente, mi permetto di fare un appello al buonsenso, perché stiamo parlando di temi molto importanti. Nessuno sta rinnegando gli accordi assunti nella Conferenza dei Capigruppo per il percorso dell'Aula, però vede, Presidente, se lei avesse la cortesia non di dare un infinito tempo a chi chiede di utilizzare il minuto, ma almeno di far finire la frase, probabilmente il clima di tensione che si percepisce in quest'Aula sarebbe minore. Pregherei quindi lei - e non il collega Romeo - di avere la cortesia di avere quella flessibilità un po' intelligente per far finire la frase a un senatore. Peraltro, al collega Romeo voglio dire un'altra cosa: può anche far finta che quello che è successo ieri non abbia rilevanza, ma a mio modo di vedere quello che è successo ieri ha rilevanza per tutti, anche per l'Assemblea del Senato. È inaccettabile, infatti, che si conducano discussioni in questa modalità e a dirlo è un Gruppo che non ha mai fatto dell'ostruzionismo una bandiera, ma quello che è accaduto ieri per me è un discrimine. Sia chiaro: non si possono picchiare i colleghi e non può avvenire una forma di violenza così grave. Dovete rendervene conto e dovete assumervi la responsabilità. È finita. Basta usare toni di questo genere.

Di conseguenza, se vogliamo essere europei, visto e considerato che fino adesso abbiamo parlato di elezioni europee, la flessibilità la do, ma la flessibilità è intransigente. *(Applausi. Commenti)*.

tramite. Il presidente Romeo ha giustamente ricordato che questo provvedimento si concluderà martedì dalle 15,30 con le dichiarazioni di voto in diretta televisiva e il voto. Mi rendo conto che voi abbiate dei problemi a mantenere il numero legale, soprattutto verso le 15,30 di giovedì e sicuramente fino a lunedì mattina o martedì vogliate andare a casa, ma non capisco però perché ci debba essere una rigidità sui tempi, avendo da oggi fino a martedì il tempo di discutere. Vorrei passare quindi a una seconda considerazione; questo disegno di legge di riforma costituzionale non prevede in ingresso nelle Aule il tempo contingentato. Mi rifiuto di vedere come una concessione il fatto che voi *(Applausi)* a maggioranza avete contingentato i tempi. E adesso devo ringraziarvi perché mi date un minuto per parlare? Ma stiamo scherzando! *(Applausi)*. Noi ci prenderemo tutto il tempo e faremo tutto quello che possiamo per dirvi fino all'ultimo secondo che state sbagliando su questa riforma e che abbiamo il diritto di parlare.

e noi per ogni emendamento faremo un nostro annuncio di voto e se non ci darete il tempo, ce lo prenderemo. Signor Presidente, prima il presidente Romeo ha detto cosa c'entra rispetto alla discussione che stiamo facendo ciò che è avvenuto ieri alla Camera e cioè calci, pugni e botte date a chi rappresenta l'opposizione. C'entra molto, Presidente, c'entra moltissimo. È il tipo di modello istituzionale che noi immaginiamo, con un Parlamento ridotto a essere residuale e quindi a non rappresentare democraticamente i cittadini e le cittadine. Eccome se c'entra quello che è arrivato ieri dalla Camera. È l'esempio davvero nefasto

1944 sono stati fucilati 60 innocenti da reparti nazisti e della Decima Mas, comandati dal più crudele, sanguinario e fascistissimo tenente Umberto Bertozzi, condannato successivamente all'ergastolo. Queste cose disonorano il Parlamento italiano e mi sarei aspettato una condanna

anch'io volevo finire il discorso di prima. La settimana scorsa vi ho detto che siete pericolosi. Non siete pericolosi solo per quello che state scrivendo nella legge, lo siete anche nei fatti, come avete dimostrato ieri.

In vent'anni ho solcato tante aule, ho fatto tanta opposizione, anzi ho fatto solo opposizione, ma non mi sono mai permesso di offendere personalmente i colleghi, di insultarli. *(Commenti.*

*(FdI)*. È impossibile. PRESIDENTE. Colleghi, per favore, facciamo parlare il collega, sia i colleghi di maggioranza che i colleghi di opposizione, per favore. È impossibile intervenire in questo contesto, è impossibile che si continui ad offendere senza che la Presidenza ci tuteli. Non sono accettabili gli interventi che ci sono stati sino ad ora; discussione leale. Gli interventi offensivi e gli insulti non sono accettabili in un'Aula del Senato e non è accettabile che proseguano così gli interventi dell'opposizione. Chiedo rispetto come senatore e credo di chiederlo a nome di tutta la maggioranza; il rispetto è mancato; si cerca la rissa continuamente, questa è la realtà.

il gesto violento, la violenza che abbiamo visto in Aula ieri, utilizzando magari termini che non sono offensivi, tipo «criminale», come la vostra presidente del Consiglio Meloni ha urlato al nostro Presidente del Consiglio e che per voi è un complimento, di fronte a un gesto fascista e squadrista che è una vergogna nelle istituzioni che state disonorando con i fatti, con riforme che attentano all'unità della Nazione e al rispetto degli equilibri dei poteri nelle istituzioni. Vergognatevi!

se un gesto simbolico e pacifico che si compie in un'Aula del Parlamento genera una reazione di violenza fisica, allora un problema ce lo dobbiamo porre, perché si stanno compromettendo la democrazia e il dialogo democratico. *(Applausi)*. Prima si è accennato all'Europa, all'Europa, che ha organizzato diversi incontri interparlamentari per parlare di dialogo democratico, di Stato di diritto, di valori condivisi. Si sta creando un problema democratico attraverso una riforma che compromette quei principi, si sta distruggendo il dialogo democratico. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a questa...

con l'intervento poc'anzi del senatore Lisei, di insulti e di attacchi, mentre noi ci stiamo riferendo al merito, parlando di un provvedimento che giudichiamo sbagliato e pericoloso per il nostro Paese. Ma, a proposito di insulti e di attacchi, lo ha già fatto ieri, con parole molto equilibrate, il senatore Manca e voglio ripeterlo io, perché ho letto il resoconto stenografico. In quest'Aula ieri il relatore Balboni ha detto (leggo dallo stenografico): la verità è che voi non perdonate all'onorevole Delmastro e all'onorevole Donzelli di aver rivelato agli italiani, che avevano diritto di saperlo, che vi stavate facendo strumentalizzare dai terroristi e dai mafiosi». *(Applausi)*. Questo è inaccettabile, caro Balboni,

Senatrice Sironi. Non ho sentito, non ho sentito. Senatrice Sironi, magari lei può ripetere cosa ha detto. *(Commenti)*.

il problema di questo provvedimento è che è pensato e strutturato dalla parte del Governo. Immagino il presidente del Consiglio Meloni sdraiata sul divano che dice: "Come posso tutelare la mia posizione? Uno, due, tre e quattro". Quello che è mancato totalmente è il punto di vista del Parlamento. I parlamentari di maggioranza non hanno lavorato a questo provvedimento, non hanno pensato di difendere il lato dei parlamentari. È puramente governativo ed è puramente autoritario. Colleghi della maggioranza - per suo tramite, Presidente - svegliatevi; svegliatevi ora, sennò sarà tardi. Signora Presidente, un intervento proprio sull'emendamento. Io continuo a esprimere, con il mio Gruppo, la contrarietà a questa visione che un parlamentare che viene indicato in sostituzione del Presidente del Consiglio eletto. Ritengo che sia sempre un tradimento dello spirito di questa legge. Se parliamo di elezione diretta del Presidente del Consiglio, quando questi, per un motivo, cessa dalla carica, non si può pensare che venga chiamato in campo un riservista. È come dire che ci sono un Presidente del Consiglio eletto e un riservista. Francamente questo non si vede da nessuna parte, in nessun sistema democratico. Quindi non capisco perché, se diamo la fiducia agli elettori e diciamo loro che possono eleggere il Presidente del Consiglio dei ministri, poi facciamo entrare dall'altra parte un riservista, che verrebbe nominato dalle forze parlamentari. Allora decidiamoci: o restiamo nella forma attuale, in cui il Presidente del Consiglio dei ministri è scelto da una composizione delle forze elette

mi rivolgo, tramite lei, ai colleghi, dopo le esternazioni che abbiamo sentito in Aula in cui il Presidente della Commissione affari costituzionali dice che è vero, quindi riconferma le sue affermazioni di ieri *(Applausi).*

caso che sia fatta così; non fate finta, siete proprio così; siete veri, siete veramente arroganti. *(Applausi)*. Davvero non avete la tenuta delle istituzioni, lo

rivolgessimo un pensiero a quell'assistente della Camera che ieri è stato picchiato ed è andato in infermeria. *(Applausi)*. Finiamo per non accorgerci di chi lavora per noi quotidianamente e ci garantisce la condizione di sicurezza. Almeno questa spero che la maggioranza abbia il coraggio di riconoscere che è stata un'aggressione.

vorrei richiamare l'attenzione del ministro Casellati su questo emendamento, che interviene - lo ricordo - sul terzo comma dell'emendamento del Governo. Non concerne quindi quei casi in cui un fatto politico determina la cessazione del rapporto di fiducia tra maggioranza e Governo, che può portare per una sola volta a un reincarico o all'incarico di un altro esponente della stessa composizione di maggioranza.

accadere, nel corso di una legislatura, troppi fatti politici che determinino la sostituzione di tanti Presidenti del Consiglio. È comprensibile. È del tutto incomprensibile il fatto che che accadimenti non politici determinino le elezioni anticipate. Vi prego di guardare quello che sta succedendo e quello che può succedere. Lo esemplifico per chi sta a casa: vince le elezioni una maggioranza che ha un Presidente del Consiglio eletto dal popolo, che dopo un mese ha un impedimento totale, come un ictus. Purtroppo succede. Viene dato un altro incarico al secondo, che muore dopo due anni. Bisogna tornare al voto. Ma perché? Qual è il motivo politico che porta a un voto per il decesso di un Presidente del Consiglio?

Com'è possibile? La Costituzione italiana, la più bella del mondo, viene rovinata dalla vostra totale incapacità. E la nostra Repubblica non può essere umiliata da un Parlamento che non accetta che si consegni un tricolore. Non è pensabile che non si accetti un tricolore.

alle ore 12,45)*. Su richiesta dei Gruppi di opposizione, sentiti i Gruppi di maggioranza, la Presidenza sospenderà la seduta, per riprendere i lavori alle ore 14.

Il senatore Enrico Borghi non era nel parapiglia, che resti agli atti. Il senatore Borghi non era inquadrato, ma era in piedi, pronto a parlare, quindi mettiamo a verbale che nulla c'entra col parapiglia creato prima. La seduta è sospesa.

su questa circostanza: oggi rivolgiamo i nostri più affettuosi auguri di buon compleanno al senatore Guidi. Riprendiamo l'esame del disegno di legge di riforma costituzionale in discussione.

dei lavori. Prima che iniziasse quel parapiglia al quale il Gruppo Italia Viva non ha partecipato - lo dico perché ho visto alcune agenzie e vorrei precisare, anche perché rimanga agli atti, che noi non abbiamo in alcun modo partecipato all'occupazione dei banchi del Governo, giusto per una piccola chiosa - volevo fare una proposta, che faccio vi sarà la discussione dell'emendamento 7.900, che è del Governo, piuttosto saliente dal punto di vista della riscrittura e del contenuto dell'articolo 7. Penso che potrebbe essere cosa utile per la decompressione dei nostri lavori che la Presidenza, *motu proprio*, concedesse cinque minuti a ciascuno dei Gruppi che ritenesse di dover intervenire, in maniera tale da consentire l'esplicazione di una questione molto rilevante e significativa (non entro neppure nel merito), affinché attorno a questa proposta, che, lo ripeto, ha fatto il Governo in via emendativa, vi possa essere un dibattito adeguato, che non sia la compressione *short* di un minuto all'interno del quale, evidentemente, come converrà con me, c'è poco più di una manifestazione d'intento. L'avrei voluto fare prima perché temevo quello che è accaduto, in una logica di decompressione, a maggior ragione lo faccio ora perché credo potrebbe essere un gesto di buona volontà da parte di tutti per consentire di concludere i nostri lavori in maniera ordinata. Grazie, Per chi è nato morto, arrivare a settantanove anni non è poca cosa, ma volevo intervenire per dire che anche oggi ci sono stati momenti di di frenesia, di creatività e anche di disagio, dall'una e dall'altra parte. Qualcuno si può preoccupare e domandarsi chissà dove andrà la democrazia. Io penso il contrario: sono tanti decenni che faccio politica e credo che, se va rigettato il concetto di chi pensa sempre di essere dalla parte della ragione criminalizzando l'altro, è anche vero che la democrazia su queste cose un po' ci ridacchia sopra. Il popolo italiano è buono, pacifico, tollerante e molto migliore di quelli che credono di non poter votare.

a una settimana dalla morte di mio fratello, quindi come sempre nella mia vita - non a caso ho fatto lo psichiatra - convivono costantemente

Posso permettermi di dire una cosa? Io stimo moltissimo il presidente Balboni, perché ha il coraggio di dire quello che pensa e quasi sempre lo condivido. Viene penalizzato per la sua sincerità, che è lo strumento più importante del fare politica. Quando voi dite "tornate indietro e ripensateci". Ripensateci anche quando penalizzate un uomo buono,

non per un qualche motivo futile, ma perché abbiamo detto che i lavori in quest'Aula non possono riprendere fino a quando non sono state pronunciate parole di ferma condanna da parte della maggioranza *(Applausi)* per le scene di inaudita violenza e di aggressione squadrista subite da un deputato già

nel vero senso della parola. Invece qui tutto tace e si vogliono riprendere i lavori come se nulla fosse, come se quella che noi abbiamo fatto fosse stata una pagliacciata. Non è stata una pagliacciata.

inclusi gli atti di violenza che possono essere stati commessi alla Camera. Ricordo che c'è un Ufficio di Presidenza alla Camera che se ne sta occupando e credo che la questione

e credo che tutti debbano averla, anche perché nell'Ufficio di Presidenza sono rappresentati tutti i Gruppi e in quella sede si prenderanno le adeguate misure nei confronti di chi si è comportato in modo scorretto e certamente la violenza è un modo scorretto di porsi. Mi permetto di dire - e infatti avrei voluto parlare anche prima che la senatrice Maiorino svolgesse il suo intervento, perché non è una novità, ma era stato detto prima il modo giusto per chiedere giustizia morale per gli episodi violenti che sono avvenuti alla Camera non è quello di violare il Regolamento del Senato, facendo un atto che non è violento, ma indubbiamente è contro il Regolamento.

C'è stato un accordo con i Capigruppo. Dovevamo riprendere i lavori ordinatamente. Senatrice Floridia, ha già parlato la sua collega di partito. Prego, senatore Malan, concluda

come dei burattini, come persone al guinzaglio e così via. Per carità, si può dire, c'è libertà, io sono il primo a difendere il diritto di dire anche queste cose, ma non è ma non è certamente il modo per affrontare gli argomenti nel merito, non è un modo per dare credibilità a quel Parlamento che giustamente difendete. Tuttavia, se permettete, lo difendiamo anche noi e ribadiamo che il Parlamento non è mortificato dal fatto di avere un Governo stabile, ma è mortificato se viene coperto di insulti e direi una storia di ieri: c'è un movimento che è nato nel disprezzo del Parlamento. Pertanto, se tutti stiamo sugli argomenti, credo che chi ci ascolta e non si stufa di sentire continue interruzioni forse capisce di più e si fa le proprie idee, senza bisogno di insulti e aggressioni verbali, men che meno di aggressioni violente, che sono sempre da condannare.

condannare tutti quanti con nettezza quanto avvenuto, affinché non ci sia silenzio e non avvenga mai più l'uso della violenza in Parlamento, in queste nostre Aule. Signora Presidente, l'occupazione dei banchi del Governo da parte delle senatrici di tutti i Gruppi di opposizione è stata

quello che è successo ieri alla Camera, contro quello che è successo due settimane fa qui in Senato, contro un clima di intimidazione in Aule che sono sacre alla libertà e al dialogo, dove si dovrebbe dare l'esempio soprattutto alle nuove generazioni. Quello che è successo ieri, signora Presidente, non è quello che è stato scritto

senatore De Cristofaro

L'emendamento del Governo è già stato esaminato in Commissione e su di esso ci siamo già espressi (la signora Ministro lo ricorderà senz'altro). È un emendamento che peraltro compare nel testo che vediamo adesso in Aula proprio perché il testo presentato dal Governo purtroppo non spiccava per chiarezza (diciamolo onestamente). Era stata proposta una sua riformulazione, che poi non è stata accolta nei lavori di Commissione come una riformulazione che potesse entrare semplicemente nel testo, perché avrebbe dato luogo alla riapertura dei termini per la presentazione dei subemendamenti; quindi si è preferito ripresentarlo in Aula, come se nulla fosse. Ma vede, signora Ministro e colleghi della maggioranza, presentare un emendamento del genere in Aula

un testo che comunque viene rimaneggiato, espressione soprattutto di un mutamento di avviso da parte del Governo proprio sull'approccio a questa riforma. originario siamo partiti infatti con la previsione che ci sarebbe stato sempre un *Premier* riservista, che sarebbe entrato in campo in ogni caso. In ogni caso in cui il Presidente del Consiglio eletto direttamente dal popolo fosse uscito di scena, era sempre prevista la possibilità dell'ingresso del riservista. Poi abbiamo fatto le audizioni e i costituzionalisti che abbiamo ascoltato hanno tutti espresso stupore per una simile ipotesi, dicendo che non si è vista da nessuna parte, che non garantiva che non garantiva la *ratio* e l'efficacia della norma, che comunque non aveva senso pensare a un Presidente del Consiglio che venisse individuato nella lista collegata. Allora il Governo, *re melius perpensa*, ha modificato il testo con gli emendamenti. Ma non era questa la versione presentata dal Governo; questa è la versione che è stata rielaborata dal presidente Pera, che infatti aveva tentato di introdurla in Commissione. Cosa voglio dire con questo? Io continuo a ritenere che il testo così non vada bene.

che è quanto previsto nel secondo comma, non mi soddisfa. Se noi investiamo i cittadini della responsabilità di eleggere direttamente il Presidente del Consiglio dei ministri, attribuiamo anche al Governo eletto in questo modo, con un Presidente che ha un'investitura diretta e popolare, la responsabilità che, se il suo mandato cessa, il Governo... mi stavo proprio avviando alle conclusioni. Su questo emendamento continuo a esprimere la nostra contrarietà, signora Ministra, e non posso che ribadirle che noi avevamo proposto un'alternativa, un testo alternativo sul quale abbiamo chiesto di ragionare, purtroppo incassando sempre un'immotivata

rappresenta il cuore della riforma, perché prevede che il Presidente del Consiglio eletto possa disporre della durata delle Camere. In questo

In questo sottoporre e rendere il Parlamento disponibile nella sua durata al Governo, noi consumiamo una trasformazione profonda della nostra democrazia. Da una democrazia pluralista fondata sul Parlamento e sulla primazia del Parlamento nei confronti dell'Esecutivo, noi stiamo, anzi voi state dando vita a un ordinamento nel quale l'Esecutivo non solo determina la composizione del Parlamento nel momento della sua nascita, ma ne dispone anche della durata. Questo è il motivo per cui abbiamo cercato e cercheremo in tutti i modi di avversare questa riforma. È una riforma che alla fine produce una mortificazione del pluralismo e della democrazia partecipativa, senza garantire in alcun modo la stabilità e la capacità di governo delle istituzioni politiche. Una centralizzazione e una verticalizzazione del potere come quella prefigurata nella riforma, oltre a non avere precedenti (non è un caso che non abbia precedenti e non abbia eguali), aprirà le porte, ancora di più di quanto già oggi non avvenga, a dinamiche demagogiche plebiscitarie che solo in apparenza consentono di esercitare una vera azione di governo dei processi economici e sociali. In realtà, più che governare i processi economici e sociali, più che mitigare le paure, più che ricondurre a unità e a razionalità le tante tensioni che sono presenti nella società, non farà altro che dividere il Paese, spaccare il Paese *(Applausi)*, accrescere le paure, accrescere la dimensione di irrazionalità. Ecco perché noi diciamo che questa riforma non soltanto mortifica e conculca la democrazia, ma non risolve nessuna delle domande di partecipazione, di legittimazione e di governo, che pure anche secondo noi sarebbe importante cercare di affrontare, ma con altri strumenti che abbiamo indicato, che è possibile percorrere e che sarebbero stati molto più efficaci e molto più rispettosi di quella che è la più grande conquista del secondo dopoguerra, ossia la democrazia pluralista pluralista e limitata, dove il potere non è concentrato in una sola figura, ma conosce invece limiti e separazioni.

molto concreto, secondo me, che questa riforma che voi proponete possa acuire ancora di più le tensioni, possa produrre elementi di lacerazione e possa farlo per di più in una democrazia come la nostra, particolarmente fragile, quella che conosciamo e che vediamo, quella in cui, come ho ripetuto ossessivamente nel corso di questi giorni, metà della popolazione nemmeno va più a votare. Quindi è una democrazia esposta a rischi di fenomeni non sempre controllabili. Da questo punto di vista, davvero condivido molto le osservazioni del senatore Giorgis. Aggiungo che questo articolo 7, che, come è stato giustamente osservato, assieme all'articolo 5 è il cuore della riforma, dimostra ancora una volta quanto sia falsa quella narrazione secondo la quale non sono toccate le prerogative del Presidente della Repubblica. È infatti del tutto evidente che, se lo scioglimento delle Camere - una delle principali prerogative che la Costituzione italiana assegna oggi alla Presidenza della Repubblica - viene di fatto sottratta al Presidente della Repubblica e attribuita al Presidente del Consiglio, ebbene, questa cosa evidentemente segna come quei poteri e quelle prerogative sono messi radicalmente in discussione. Ne discuteremo ancora, ma davvero almeno non si utilizzi più questo argomento, secondo il quale questa riforma è soltanto un intervento chirurgico che non scombussola l'ossatura della Costituzione italiana. Lo fa invece fino in fondo e lo fa a partire da uno dei punti più importanti: le prerogative e i poteri del Presidente della Repubblica di questo Paese.

Mi viene in mente una metafora calcistica, che forse è di facile comprensione: stiamo vivendo una situazione ipotetica in cui uno dei giocatori a un certo punto decide che il gioco si ferma, prende la palla, lascia il campo e se ne va. Questa è prerogativa di un arbitro, non di un giocatore. Quindi, noi stiamo dicendo che il Presidente del Consiglio si arroga il ruolo dell'arbitro e non è così, perché sta da una parte. *(Applausi)* Inoltre, c'è un'altra incongruenza palese in uno dei casi che viene annoverato, cioè quando il Presidente del Consiglio eletto decida di non dimettersi, ma chiede che il Presidente della Repubblica gli conferisca l'incarico di formare il Governo. È chiaro che questa è l'ipotesi che si verificherebbe nel momento in cui il Presidente del Consiglio non può più fare conto sulla propria maggioranza. Quindi, voi, paradossalmente, state istituzionalizzando il ribaltone; fondamentalmente il Presidente del Consiglio può chiedere l'appoggio di forze politiche diverse da quelle attraverso il cui consenso è diventato Presidente del Consiglio. Sta tradendo il voto degli elettori. Ci sono tanti aspetti gravissimi e incongruenti in questa riforma, per cui caldeggio fortemente uno *stop* e una riflessione tutti insieme.

In questi giorni ho sentito il ministro Alberti Casellati, che, rivolgendosi all'opposizione, ha detto sostanzialmente che non ci sono state proposte alternative e che se ci fossero state proposte alternative fatte dalle opposizioni, si sarebbe aperta una fase diversa di dialogo.

Sul metodo abbiamo detto che questo non è un clima nel quale procedere alla riforma costituzionale. Mi dispiace, ma quello che succede in tutti e due i rami del Parlamento dimostra che che avevamo ragione, perché questo non è un clima nel quale si può fare una condivisione di una riforma costituzionale. Nel merito, signora Ministro, noi, come Azione e lei lo sa, avevamo proposto un modello alternativo al premierato, che è quello del cancellierato alla tedesca. anche su questo emendamento noi avevamo proposto la mozione di sfiducia costruttiva, proprio per dimostrare che il rapporto deve essere sempre tra il Parlamento e la maggioranza con delle modalità che contengano la funzione parlamentare, senza obbligare il Presidente allo scioglimento. Quindi, non è vero che non ci sono state modalità diverse, sia nel metodo che nel merito. Se non sono state accolte e non state accettate è perché - continuo a ribadirlo la riforma confonde un punto vero per tutti, cioè la stabilità del Governo, con un punto vero solo per questa maggioranza, cioè la stabilità del Capo del Governo. Sono due cose diverse e noi rivendichiamo il nostro posizionamento, sul quale chiediamo ancora una volta di esprimere un giudizio e anche - così concludo stando nei miei tempi, Presidente - rivendicando che c'è un modo che noi interpretiamo, non perché non riconosciamo l'ostruzionismo e la modalità usata dal resto dell'opposizione, ma se chiediamo agli italiani di rispettare la riforma costituzionale, io ritengo che sia doveroso anche che noi stessi rispettiamo il Regolamento del Parlamento tutte le modalità con le quali si può stare in Aula ad esprimere fortemente il proprio dissenso, ma anche con delle modalità diverse.

Signor Presidente, si tratta di un ordine del giorno già votato in Commissione. in seguito alla trasformazione di un emendamento del presidente Pera. Quindi, confermo il parere favorevole.

lascio agli atti che noi stiamo qui discutendo di una riforma costituzionale che nasce dal Governo, ma è nella piena disponibilità del Senato. Se la maggioranza affronta un tema così delicato attraverso un ordine del giorno, io mi chiedo se

a chi è rivolto l'ordine del giorno. A chi ci stiamo rivolgendo? A chi vi state rivolgendo? A chi state chiedendo di prendere un impegno? Stiamo riformando la Costituzione e voi, su un aspetto decisivo, impegnate l'Assemblea a chiedere a chiedere a chi? Di impegnarsi a fare cosa? Un po' di serietà, per cortesia.

l'emendamento all'ordine del giorno, ma, alla domanda specifica, a chi si rivolge questo ordine del giorno, rispondo con un'altra domanda? A chi si rivolse l'ordine del giorno Perassi in Assemblea costituente? *(Applausi)*.

riferito a lei, ma non ho sentito. *(Commenti)*. Invito i colleghi della maggioranza

Vorrei fare due considerazioni molto rapide, la prima di carattere formale, la seconda di carattere sostanziale. Io penso che sia giusto che l'Aula sappia che questo ordine del giorno è frutto di un precario equilibrio raggiunto all'interno della maggioranza, perché a questo ordine del giorno si è pervenuti dopo uno scontro tra le forze di maggioranza all'interno della Commissione. Tale scontro ha provocato anche una interruzione dei lavori della Commissione, il ritiro dell'emendamento presentato dal presidente Pera e la formulazione di questo ordine del giorno. Quindi, si è arrivati a manifestare su un punto specifico quella tensione di natura politica, alla quale io facevo riferimento anche nei giorni scorsi, che tanto aveva provocato la reazione della ministra Alberti Casellati, relativa ad uno scontro interno alla maggioranza tra le visioni di chi ritiene che sullo sfondo dell'equilibrio istituzionale vi debba essere un doppio turno con ballottaggio e chi, invece, all'interno della maggioranza ritiene che la legge elettorale debba circoscrivere, all'interno di un unico turno con trascinamento, la chiusura di questa partita. Questo ordine del giorno è frutto di uno scontro interno alla maggioranza e, nel merito, pretende di bipartitizzare il nostro sistema e noi non possiamo accettare che con un ordine del giorno si tenti una forzatura di questa natura, perché l'intento, che naturalmente può essere l'intento, che naturalmente può essere apprezzabile dal punto di vista della proposta, di imporre il modello Westminster alla Repubblica italiana, modifica in senso strutturale e profondo il sistema della rappresentanza nel nostro Paese. Questo non si può fare con un ordine del giorno. per dichiarare il voto contrario. In questo caso sono molto d'accordo con le considerazioni che faceva adesso il senatore Borghi. In Commissione, quando ne parlammo, per motivare il mio voto contrario dissi che ero contro l'individuazione

a una misura che obiettivamente stravolgerebbe radicalmente il sistema politico, non solo introducendo il premierato, quindi l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma di fatto operando una novità culturale epocale in questo Paese, quindi assimilando l'Italia molto di più a quei Paesi non semplicemente bipolaristi, bipolaristi, ma bipartitici, quelli per l'appunto tipici dei sistemi anglosassoni come il Regno Unito e gli Stati Uniti, che non lo sono neanche più, peraltro, perché i fatti che sono accaduti in questi anni dimostrano come quel bipartitismo evidentemente non regge più alla luce dei cambiamenti che sono intercorsi nella società.

evidenzia alcuni elementi di differenza molto seri che ci sono tra le forze di maggioranza e che mi porta a dire che è proprio la dimostrazione della poca serietà con cui è stata trattata Signora Presidente, parto da quello che diceva il senatore De Cristofaro, ossia che stiamo lavorando in un clima surreale. Vorrei fare un paragone. Quando un chirurgo deve intervenire su un organo vitale - sul cuore, sul fegato - aspetta che le condizioni di quel paziente siano quantomeno tranquille e stabili e non ci sia un'infezione in corso. Così, quando si interviene su una riforma così importante, - anzi, su due riforme, perché in parallelo stiamo intervenendo anche con l'autonomia differenziata alla Camera -, quando si interviene sul cuore della Costituzione, su riforme che segneranno per sempre il futuro di questo Paese, non solo si dovrebbe aspettare una condizione di stabilità, di pace sociale che in questo momento assolutamente non c'è, ma quantomeno un clima sereno per lavorare in Parlamento. *(Applausi)*. Come è possibile che pretendiate che qui oggi lavoriamo in maniera serena, se non siete nemmeno riusciti a condannare chiaramente l'attacco squadrista che c'è stato alla Camera?

visto che abbiamo superato l'articolo 7 e lo abbiamo approvato, volevo intervenire per un minuto soltanto per ringraziare la Ministra dell'emendamento appena approvato appena approvato perché risolve una delle più grandi brutture presenti in questa riforma costituzionale, anche se ne restano tante. Tale misura ha tolto quella frase che veramente era uno sfregio alla Presidenza della Repubblica. Prima si diceva che in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, costui può proporre lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone. Quindi, fino a cinque minuti fa, avevamo una Costituzione nella quale il Presidente del Consiglio propone e il Presidente della Repubblica dispone. Ora, più o meno la sostanza resta sempre quella, ma almeno in questo emendamento del Governo avete tolto questa frase che era veramente orribile.

a mio avviso, ancora qualche parola sulla questione di cui abbiamo discusso prima sullo Statuto dell'opposizione e lo faccio dichiarando il mio voto favorevole all'emendamento 7.0.1001. Il motivo per cui noi ci siamo trovati di fronte a questa farsa dell'ordine del giorno, vorrei ricordarlo, è duplice: da una parte, c'è stata una lite interna alla maggioranza perché l'emendamento presentato dal senatore Pera prefigurava una situazione di bipartitismo e, quindi, di dominio di un partito all'interno della coalizione e ovviamente le componenti minoritarie della maggioranza, maggioranza, dopo un lungo conclave, hanno bocciato l'idea di far andare avanti questo emendamento e l'hanno trasformato in un ordine del giorno privo di forza e destinato a nascondere questo fatto.

per dichiarazione di voto. rientra nell'esigenza che abbiamo tentato di riproporre più volte di omogeneità. In particolare, questo emendamento propone che il Primo Ministro possa revocare con proprio decreto i Ministri. È di tutta evidenza che se si va nella direzione dell'elezione diretta del Primo Ministro, questo debba avere la responsabilità piena dell'Esecutivo anche in termini di individuazione dei Ministri e di revoca nel momento in cui essi non sono più funzionali alla propria attività. È quello che accade negli altri casi di elezione diretta nel nostro Paese, cioè nel caso dell'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di Regione. Anche su questo siete riusciti invece a costruire un papocchio, un imbroglio, una confusione.

con chi propone emendamenti di merito, per spiegarci semplicemente perché un emendamento come questo non può essere accolto e non va nella direzione di garantire la stabilità

al solito, ci imbattiamo in un testo in cui la maggioranza si fa vanto di aver fatto interventi in punta di penna, come se questo fosse garanzia di una riforma efficace e soprattutto puntuale, laddove invece le modifiche che vengono proposte e sulle quali ci stiamo confrontando sono parziali e spesso non considerano che,

Signora Presidente, vorrei sottolineare quanto sia avvilente ascoltare i colleghi dell'opposizione fare proposte nel merito e,

spiegare il motivo per cui, viceversa, state sostenendo la bontà delle vostre deduzioni. In questo caso, invece, le critiche fondate vengono lasciate cadere e si passa direttamente al voto. Se non è autoritarismo questo, ditemelo voi

Signora Presidente, questi sono gli ultimi emendamenti all'articolo 7, pertanto ci avviciniamo ad un voto importante su un articolo che riguarda specificatamente il ruolo del Parlamento, e quindi di noi senatori e senatrici, rispetto alla nascita e alla morte di ogni Governo. È quindi l'ultima occasione che abbiamo per riflettere ancora su quello che stiamo andando a votare, per riaprire una discussione, anche con i colleghi di maggioranza, su una questione che ci riguarda direttamente, non solo nel nostro ruolo attuale, ma in quello che consegneremo a chi verrà in queste Aule dopo di noi. Per suo tramite, signora Presidente, chiedo quindi ai colleghi di maggioranza di cederci una parte del loro tempo residuo per riaprire la discussione, altrimenti la votazione di questo articolo e del successivo perderà di *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, ci stavamo confrontando con il collega senatore Marton sul motivo di questa disomogeneità e giustamente il collega mi faceva presente un aspetto che vorrei riportare all'Assemblea, perché a mio giudizio è la verità. Perché questa maggioranza, da una parte, consente l'elezione diretta del Primo Ministro, dall'altra, lo imprigiona nella impossibilità di scegliere i Ministri? Lo fa perché vuole mantenere la ragnatela del condizionamento dei partiti nei confronti del Primo Ministro, qualcosa del seguente tipo: è vero, vieni eletto dagli italiani, ma poi devi passare dalle nostre forche caudine, per cui non ti sognare di mettere in discussione la revoca di un nostro Ministro. Voi ve la immaginate Giorgia Meloni revocare il mandato a Matteo Salvini? È evidente che quindi si vuole costruire una ragnatela nella quale solo nominalmente il *Premier* ha più poteri, ma in realtà sarà un *Premier* imprigionato.

Peraltro, come lui sa, non essendo d'accordo con l'elezione diretta, non sono nemmeno d'accordo con il potere di revoca e di nomina, e anzi rivendico il fatto che nella Costituzione italiana il Presidente del Consiglio (che si chiama così e non si chiama Primo Ministro) sia un *primus inter pares*, esattamente come era un *primus inter pares* nazionale per marcare una totale discontinuità rispetto agli anni precedenti. Non fu un caso che era un *primus inter pares*; era così perché quella era stata la forma che aveva scelto il Comitato di liberazione nazionale, esattamente per segnare tutta la discontinuità possibile

visto che la maggioranza non l'ha saputo fare e mi dispiace molto, perché ho stima del senatore Malan, ma è stato incapace di dire ciò che è evidente dalle immagini, che un'aggressione è un'aggressione e non è una rissa e che la violenza va condannata. *(Applausi)*. Lo faccio io, da insegnante, e lo faccio come MoVimento 5 Stelle. Lo dico ai ragazzi fuori: quello che avete visto ieri è veramente incredibile, è una scena da condannare e sono certa che la condanniamo tutti. Lo diciamo noi, visto che la maggioranza è stata incapace di dirlo. Presidente, noi riteniamo che sia veramente impossibile fare finta di niente. Noi odiamo gli indifferenti. Senatore Malan, prima di occupare pacificamente i banchi del Governo, per un'ora abbiamo fatto interventi dicendo e chiedendo che la maggioranza condannasse quell'atto di violenza. E non lo avete fatto. Quindi noi riteniamo che in questa situazione sia veramente impossibile continuare i lavori. Lo dico ai ragazzi fuori: scusate davvero per le scene indecenti che avete visto.

senatore Giorgis che è tutt'altro che irrilevante. Vorrei che il Governo o il relatore spiegassero a tutti i senatori, e a chi eventualmente sta seguendo i lavori, che cosa accadrà se

a seguito di una consultazione popolare, perché è chiaro che i due terzi non li raggiungerete. Immaginiamo che non venga prontamente approvata questa fantomatica legge elettorale, di cui al momento mi sembra non abbiate la più pallida idea di come definire. Che cosa accadrà al nostro Paese? Nel Nel momento in cui la riforma venisse approvata, dal punto di vista delle fonti costituzionali entrerebbe in vigore, quindi ci troveremmo ad avere un ordinamento costituzionale che, secondo quanto prevede la norma transitoria, non entra in vigore, perché entra in vigore soltanto dopo che verrà approvata la legge elettorale. Ma se la legge elettorale non venisse prontamente approvata, noi ci troveremmo - e questa è la domanda che faccio al relatore e al Governo - in una situazione di sospensione costituzionale, con un Parlamento con dei cittadini che si sono pronunciati per una Costituzione che però non è applicabile e non entra in vigore, perché la norma transitoria ne subordina l'efficacia all'approvazione della legge elettorale. Poi avremmo una Costituzione invece che che è stata abrogata dalla nuova Costituzione, ma che non si può più applicare. Vi rendete conto di cosa vuol dire produrre un tale effetto di incertezza sul piano delle fonti e su quello della tenuta costituzionale e sull'ordinamento? Questo

premesso che è sempre meglio discutere e fare opposizione restando in Aula che non uscendo. Forse una risposta potrebbe essere quella che si voglia approvare il disegno di legge magari con entrambe le letture, ma non è detto che che si voglia davvero rendere operativa la riforma costituzionale, perché si sa perfettamente che ci potrebbe essere un *referendum* e magari si vuole posticipare quel *referendum* alle prossime elezioni. elezioni. Probabilmente, una delle risposte possibili del perché non abbiamo quello che vogliamo, cioè la contezza di qual è la legge elettorale, è perché c'è una mossa molto politica e tattica che ha a che fare con il rinnovare la volontà degli elettori. È come se la volontà degli elettori potesse essere legittima solo nel momento in cui si esprime sulla Presidenza del Consiglio o sul premierato e non fosse altrettanto legittima quando chiede che i rappresentanti del popolo siano i parlamentari.

mi scusi, ma vi rendete conto di cosa vuol dire sottoporre al voto dei cittadini un testo, la cui applicabilità dipende da una legge che i cittadini stessi probabilmente non conosceranno e che non entrerà in vigore neanche se i cittadini si dovessero pronunciare a favore? Vi rendete conto di quale precedente state creando nel nostro ordinamento costituzionale?

Se gli emendamenti sono proposti da coloro che non sono in Aula, si votano o decadono? Perché, se decadono, probabilmente avrebbe senso che i colleghi tornassero in Aula per difenderli.

siano proprio indicative di come non si sia voluto cercare in alcun modo, in tutti questi mesi, già in Commissione e adesso in Aula, una possibile sintesi tra le forze politiche in questo Parlamento su una cosa così importante e così seria come la Costituzione italiana. Si è scelta un'altra strada, si è scelto di andare avanti a colpi di maggioranza, senza ascoltare le opposizioni. Peraltro, lo si è fatto anche generando un clima in quest'Aula e in quell'altro ramo del Parlamento che penso sia particolarmente negativo per questo Paese, che rischia di accendere anche lacerazioni di cui il Paese certamente non ha bisogno. Credo che abbiano fatto molto bene le forze di opposizione a ritrovarsi, come faranno martedì prossimo, in piazza a convocare una manifestazione. Saremo lì, ci vedremo in quella piazza, in una piazza che denuncerà quello che è accaduto in questi due rami del Parlamento in questi giorni, il clima che si è determinato, le continue forzature e che dirà nella maniera più chiara possibile che a partire da quella piazza difenderemo non soltanto in queste Aule parlamentari, ma innanzitutto tra i cittadini di questo Paese, la nostra Costituzione repubblicana. Nessuno pensi che basti semplicemente un voto di quest'Aula per cambiare la Costituzione, per stravolgerla. Fortunatamente ci sarà un *referendum* e sono assolutamente convinto

Presidente, siamo arrivati con grande difficoltà sin qui. Voglio lasciarlo agli atti per i colleghi della maggioranza che minimizzano, qualcuno ironizza anche, non capendo o non dando il giusto valore valore al deliberato che verrà fuori da queste sedute. L'ho sottolineato più volte nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e lo ribadisco qui in Aula. Il presidente Malan, il presidente Romeo, il presidente Gasparri

il lavoro faticosissimo fatto da tutte le colleghe e i colleghi della Commissione affari costituzionali e da tutti i colleghi e le colleghe in Aula, democraticamente rispettoso delle regole, ci ha portati fin qui. Presidente Pera, lei più volte ha richiamato, nei momenti più difficili del nostro dibattito, alcuni passaggi della Costituente. Glielo chiedo per la sua storia, per la storia di quest'Assemblea: quando lo fa, se le capiterà, la prossima volta ci aggiunga anche i nomi di De Nicola, De Gasperi, Terracini e Grassi *(Applausi)*, perché danno il senso il senso di quelle firme sotto la nostra Carta costituzionale e danno ancora di più il senso della responsabilità che vi state assumendo per modificare la Costituzione. Quelle firme sono un pezzo della nostra storia. Non vi faccio le biografie dei singoli, ma non a caso c'erano

il tentativo di avere delle possibilità sempre aperte. Come ci siamo detti più volte e la signora Ministra sa, la democrazia non è data, è una sperimentazione continua. Le possibilità aperte che ci dà la nostra Carta costituzionale e che ci sono ancora anche alle modifiche, sono connesse alle trasformazioni sociali. Evoluzioni sociali, presidente Pera, non involuzioni sociali. Ci preoccupano le cose che stiamo leggendo oggi a margine del G7. Se infatti la modifica della Costituzione intercetta anche quelle involuzioni sociali - questa è la sensazione che abbiamo - facciamo molto male al nostro Paese.

comune. Tale consenso deve essere sempre e solo ritenuto prossimo al bene sociale, non al bene di una forza politica o di due forze politiche che fanno uno scambio. Signora Presidente,

Noi saremo in Parlamento e faremo sentire rispettosamente la nostra voce, ma saremo anche e soprattutto in piazza con tutte le opposizioni e con tutte le persone che vorranno... questa battaglia che è soprattutto culturale e poi anche politica, il senso della nostra dignità collettiva. Signor Presidente, conclusione, che noi ci fermiamo qui, non parteciperemo simbolicamente all'ultimo voto perché riteniamo che le forzature che ci sono state rispetto ai tempi e alle prerogative delle opposizioni si potevano evitare.

Senatrice Malpezzi, se vuole venire al posto mio la invito, ma l'ho vista e l'ho ripresa. Senatore Boccia, solo per mettere agli atti, a proposito dei tempi, che questo è il sesto minuto. Ma prego, vada pure avanti.

Signora Presidente, concludo denunciando lo scambio che c'è stato - ed è stato plastico soprattutto a Montecitorio nelle scorse ore - tra le due forze politiche. Non a caso dico due forze politiche perché ieri Forza Italia, che è un partito che lei conosce bene, aveva una discussione interna molto evidente. Avevamo ad un certo punto preso atto della richiesta di voto contrario del presidente della Regione Calabria, Occhiuto, che non è un deputato, ma è un autorevole esponente

per votare a Montecitorio spaccherà il Paese. Siamo certi di una cosa: sul premierato avremo gli strumenti che i Padri costituenti ci hanno dato, a partire dal *referendum*, sull'autonomia faremo di tutto per fermarvi a Montecitorio e martedì in piazza, e se non lo farete, raccoglieremo le firme perché anche lì deciderà il popolo italiano.

abbiamo detto più volte, che quando si fa il confronto fra il numero di sedute occorse nel 2016 e quelle di questa legislatura... A quanto pare qualcuno non gradisce ricordare la realtà. Vorrei ricordare che all'epoca il Regolamento prevedeva che ci fossero due sedute, se non addirittura tre, quando c'è anche la seduta notturna. *(Commenti)*. Dal 2018 invece c'è una sola seduta. Noto lo stile del senatore Sensi che, dopo aver detto cose molto peggiori, oggi mi dice di fare il contabile perché sto tentando di ristabilire la verità. Aggiungo che una collega del MoVimento 5 Stelle ha detto che l'atmosfera non è tale da poter continuare. Faccio notare che l'atmosfera non è tale da poter continuare per decisione dell'opposizione, che ha deciso di fare degli interventi *(Applausi),* occupare i banchi del Governo, occupare il banco del Presidente del Senato. *(Applausi)*. Certamente il clima è quello, ma non si può creare un clima…

costituì nel 1956, dopo che una legge approvata dal Parlamento ha stabilito come attuarla. Ricordo che le Regioni a statuto ordinario, stabilite dalla Costituzione nel 1948, hanno iniziato a funzionare nel 1970, dopo che una legge ordinaria del Parlamento ha stabilito le modalità di elezione. *(Applausi)*. Per cui non stiamo facendo nulla di nuovo e ricordo che nella Costituzione c'è anche l'articolo 138, che ne stabilisce le modalità di cambiamento; potevano scriverlo in altro modo, potevano mettere dei vincoli più pesanti, come ci sono, per esempio, negli Stati Uniti d'America; lo hanno stabilito in questo modo sempre quegli stessi Padri costituenti, tra i quali l'onorevole Terracini era tra quanti erano contrari all'istituzione dei senatori a vita. Anche le sue opinioni erano rispettabili, come lo sono anche le nostre.

che la maggioranza non possa attuare il suo programma elettorale. *(Applausi)*. Come abbiamo detto più volte, noi siamo al ventesimo mese della legislatura - io l'ho detto in vari interventi e lo ripeteremo

ribattere a ogni astrusità che viene detta in quest'Aula sul fascismo, sulle dittature e quant'altro. Abbiamo sentito un elenco di argomenti ridicoli e non un dibattito vero di merito, che il ministro Alberti Casellati ha aperto mesi e mesi fa, incontrando i Gruppi parlamentari e le forze politiche, tant'è vero che il centrodestra, come è stato detto - e lo si ripeterà -, era partito da un programma più ambizioso di presidenzialismo e ha ritenuto il premierato, con tutta la salvaguardia dei poteri e delle funzioni del Presidente della Repubblica, già una forma di adeguamento a un pensiero più condivisibile nel Parlamento. Dopodiché la citata descrizione fantascientifica viene fatta da chi è abituato a prendere i Presidenti del Consiglio nei giochi di Palazzo: questo avete fatto per tutta la vita con Enrico Letta, con Paolo Gentiloni, con Matteo Renzi, che non vedo darci lezioni. Ho la scatola di babbi pronta per lui, così non deve andare nemmeno all'autogrill quando verrà. È vuota, come le urne per Renzi del resto. Ci siamo presi settimane di lezioni, elenchi infiniti di sedute e poi si abbandonano i lavori. Devo anche esprimere un rammarico (l'ho già fatto in privato al senatore Patuanelli e al senatore Boccia): ci meritavamo una contestazione migliore. Le bandiere tricolori dei vostri colleghi alla Camera sono meglio di quei cartoncini malmessi. Se dovete sventolare il tricolore, fatelo bene. Contestateci bene e non con quattro pezzi di carta. Buon viaggio verso il *week-end* e fate presto che a Fiumicino c'è traffico, l'aereo aspetta.

*(Misto-Az-RE)*. A tutti quelli che mancano, perché credo che sia giusto fare, nonostante tutto, la battaglia parlamentare in tutti i modi che l'opposizione ha a disposizione. Sono legittimi quelli in cui l'opposizione abbandona l'Aula e sono legittimi quelli in cui l'opposizione rimane qui. Però, Presidente, non posso non interloquire con il collega Malan (per il suo tramite), se ho trenta secondi, visto che tanto ormai siamo pochi, quindi possiamo intervenire.

che le riforme siano ragionate, condivise, siano fatte in un clima diverso da quello nel quale purtroppo ci stiamo muovendo. L'idea che si possa fare una riforma costituzionale, ovviamente condizionata dal fatto che poi entrerà in vigore successivamente il piano, è la conferma di quanto io prima dicevo, cioè che voi volete portare a casa il punto del premierato, ma volete prima che si vada alle prossime elezioni, in modo che il voto elettorale possa legittimare quello che voi state dicendo. È la conferma di un'opinione che discutevamo con il collega e che probabilmente nelle sue parole trova la prova del nove.

un'occasione mancata rispetto a quello che è accaduto. Vede, signora Presidente, la memoria non può non tornare, visto che stiamo parlando della riforma strutturale della nostra Costituzione, a quando, nel gennaio del 1947, si ruppe l'intesa tripartita che consentiva il Governo del Paese e che aveva assicurato, fino a quel momento, l'espressione di un quadro politico omogeneo nei lavori dell'Assemblea costituente. Fu una rottura profonda e pesante, che vide da un lato la Democrazia Cristiana e i partiti laici e dall'altro il Partito Comunista e il Partito Socialista. I lavori dell'Assemblea costituente erano divisi nel seguente modo. Alla mattina il Parlamento, in forma monocamerale nella circostanza, si riuniva per gli affari di Governo e volavano i calamai, come ci dicono le cronache dell'epoca; c'erano risse, anche allora, e c'era fortissima tensione. Poi, al pomeriggio, ci si riuniva per discutere del testo della Costituzione e le stesse forze politiche, le stesse persone fisiche che alla mattina si erano così fortemente contrastate trovavano un punto di convergenza e di condivisione, perché avevano ben chiaro quale fosse l'elemento della partita, quale fosse la posta in gioco, quale fosse il valore intimo del senso più profondo della Carta costituzionale. Non possiamo che esprimere quindi il nostro rammarico per il modo con il quale da ambi i lati - me lo faccia dire - non si è voluto fin dall'inizio costruire uno spirito costituente, uno spirito di reciproco ascolto, uno sforzo di condivisione e di comprensione delle ragioni dell'altro. Anche i toni, le parole e le modalità che da ultimo abbiamo sentito (penso ai toni dileggianti e anche bulleschi del senatore Gasparri di pochi minuti fa) dimostrano evidentemente quale fosse il vero e il reale intento di questa maggioranza. però non diamo soddisfazione a chi punta tutto sulla logica del «o di qua o di là», alla logica del «o la va o la spacca», alla dimensione di un finto bipolarismo di contrapposizione che vede poi, dentro questo gioco degli specchi, i *leader* dei principali schieramenti, che oggi qui ritengono di doversi confrontare e scontrare, chiamarsi il giorno dopo delle elezioni per farsi reciprocamente i complimenti fra loro *(Applausi)*, in gioco teatrale dal quale la Costituzione dev'essere sottratta. Noi saremo qui, faremo fino in fondo il nostro dovere di opposizione che vuole entrare nel merito e portare le proprie opinioni e che rifugge una dimensione

e nell'ultima votazione mi consenta di dire che i simboli in democrazia e il rispetto delle regole hanno un valore e ognuno li rispetta secondo la propria coscienza e il proprio modo di fare politica. Ognuno giustamente pensa di interpretare il modo di fare opposizione come lo ritiene più opportuno. Io non giudico gli altri, ma ho la mia modalità. Tramite lei, signora Presidente, rispondo al collega Lisei che diceva: io sono stato all'opposizione e sono stato in maggioranza; quando sono stato all'opposizione, ho rispettato le regole della democrazia. Corretto? Io ero in maggioranza nelle occasioni in cui il senatore Lisei era all'opposizione e credo che anche la maggioranza abbia la responsabilità di consentire all'opposizione di farla. Ci sono queste due modalità, perché nella vita si può essere sia all'opposizione, sia in maggioranza, ma se non rispettiamo le regole se non rispettiamo le regole del nostro convivere civile, le norme previste nei Regolamenti, come possiamo chiedere di rispettare la più ampia delle leggi che ci tiene tutti insieme, cioè la nostra Costituzione? In questo senso, Presidente, la mia presenza qui e la presenza del partito che rappresento, cioè Azione, non vuole essere un elemento di collaborazione nei confronti della maggioranza, ma semplicemente di rispetto nei confronti delle regole e di questa Istituzione.

in questo che è l'ultimo intervento prima della prossima settimana, quando ci saranno le dichiarazioni di voto. È un momento, a mio avviso, importantissimo. Non avrei mai voluto consegnare l'esempio a mia figlia di non essere presente in Aula e di non prendere la parola e non difendere fino all'ultimo la nostra visione, il nostro progetto e il disegno che anche noi avevamo presentato. La nostra presenza qui testimonia che l'impegno si difende sul campo fino all'ultimo. Io la penso così, così la pensa il mio Gruppo e siamo qui proprio per questo motivo. mi metto anche nei panni della maggioranza. È il vostro programma di Governo, quello per il quale siete stati eletti e avete nuovamente investito le urne di una richiesta di fiducia. Avete ragione voi: lo dovete portare avanti, anche se ricordo che il vostro programma era più orientato a fare il presidenzialismo che non questa riforma, che è un po' un ibrido, una novità assoluta. Avete quindi una grande responsabilità: la maggioranza ha una grande responsabilità; il Governo ha una grande responsabilità. che ci fosse più capacità, però, anche di dialogare con le opposizioni, soprattutto con l'unica forza dell'opposizione che si è confrontata, o almeno si è messa a disposizione veramente - per farlo - per confrontarsi sul testo e migliorarlo, perché, a nostro avviso, era un testo che andava migliorato. Per questo dico che è un momento fondamentale, perché non stiamo discutendo di un provvedimento qualsiasi, ma di una riforma costituzionale, che andrà chiaramente alla verifica del voto popolare

Si è così esaurito l'esame degli emendamenti. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, le dichiarazioni di voto finali avranno luogo nella seduta di martedì prossimo, 18 giugno, a partire dalle ore 15,30.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

Modifiche alla parte seconda della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

Grazie,